Comunico inoltre che, in data odierna, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze:* «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia»

La seduta è tolta